Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo prevedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Campania a seguito dell'opzione derivante da una situazione di incompatibilità del senatore Vincenzo Cuomo per la carica di sindaco della città di Portici, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Lucia Esposito. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Lucia Esposito. *(Applausi)*. Avverto che da oggi decorre nei confronti della nuova proclamata il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

giovedì scorso. Il senatore Giovanardi è intervenuto trattando la questione delle attività circensi

che prevede l'eliminazione graduale delle attività che fanno uso di animali all'interno del circo. Come sanno i membri della Commissione, abbiamo cercato di trovare una soluzione che potesse essere abbastanza di equilibrio e crediamo comunque che quella individuata abbiamo inserito all'interno del provvedimento molte misure che prevedono strumenti di incentivazione e misure di semplificazione amministrativa,

nei confronti del mondo del circo, che è storicamente consolidato e fa parte della nostra tradizione e cultura e della cultura dello spettacolo. E questo principio di delega si inserisce in un quadro legislativo che da tempo incentiva le attività senza l'utilizzo di animali proprie un circo contemporaneo. Vi è, quindi, un processo di riconversione già avviato e il provvedimento si inserisce all'interno di siffatto filone.

di derivazione internazionale ed europea, le quali pongono limiti e condizioni per la detenzione e l'utilizzo degli animali in via di estinzione, selvatici e pericolosi.

eliminazione» - la quale sarà collegata alle particolari cautele da seguire per garantire il benessere degli animali, sostenendo gli oneri, non indifferenti, per l'idonea collocazione degli animali, che in molti casi sono esemplari di specie in via di estinzione e nati in cattività. E di questo si deve tenere conto, ossia del massimo dell'equilibrio e del rispetto del processo complessivo di graduale superamento di una tale modalità

che hanno a cuore il benessere degli animali con cui lavorano. Per questo, pur comprendendo le sue ragioni, senatore Giovanardi, la invito a riconsiderare, sulla base di queste mie considerazioni, una posizione che, mettendosi in una logica di contrapposizione assoluta, sicuramente non aiuta il processo, che deve essere molto graduale e deve dare spazio e tempo al mondo del circo e consentire agli animali, che sono la nostra prima preoccupazione,

chiaro a tutti. Tutto il settore dello spettacolo è disciplinato con decreti-legge convertiti, come abbiamo già ricordato. Le risorse, in un transitorio perenne, sono assegnate con decreti non aventi natura regolamentare, che fondano le loro basi normative su leggi risalenti nel tempo. Pertanto, se c'è un minimo di soddisfazione,

che non ha cittadinanza nelle norme. Il disagio di artisti italiani di fama internazionale come Roberto Bolle - è stato citato dalla collega Montevecchi - può trovare riscontro in quest'Aula. Noi abbiamo finalmente parlato di danza; abbiamo dato cittadinanza alla danza anche in quest'Aula.

il testo in realtà non modifica il quadro, ma prosegue con energia su una strada segnata da anni, e da ultimo con l'intervento d'urgenza nel decreto sugli enti locali, convertito nella legge n. 160 del 2016. Le risorse destinate in quota Fondo sono oggi poco più di 180 milioni di euro, a cui si aggiungono 20 milioni straordinari assegnati dalla legge di bilancio per il 2017 e anche dal milleproroghe del 2017. Si tratta quindi di interventi importanti e chi ha detto, anche in questo dibattito, che non c'è alcuna discontinuità

sull'accentramento di poteri in capo al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. A questo proposito, colleghi, vi suggerisco una diversa lettura del disegno di legge. legge. La previsione di un organismo - ci si riferisce al consiglio superiore dello spettacolo - con rappresentanti di diverse anime, delle categorie e di tutte le varie arti con il compito di valutare gli effetti delle misure previste sullo sviluppo del settore, dovrebbe essere una garanzia di dialogo

per puntare a una logica di sostanza, dove, in presenza di poteri marcati di indirizzo politico, ma anche di luoghi di dialogo e verifica dei risultati, si possano maturare scelte adeguate per lo sviluppo del sistema. Ci sarà un coinvolgimento di tutti i soggetti dello spettacolo e questo mi sembra un elemento un elemento molto importante e anche molto significativo del provvedimento. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Tosato,

Nel solco dell'esperienza degli ultimi anni, i regolamenti di delegificazione e i nuovi criteri di riparto del FUS per le fondazioni seguono una logica volta a distinguere tra le realtà virtuose e quelle problematiche

patrimonio storico della Nazione, e lo sviluppo complessivo delle attività culturali, che si coniugano bene anche ai luoghi dell'arte e che, attraverso gli spettacoli, possono avere una valorizzazione maggiore. È uno dei cavalli di battaglia del ministro Franceschini, che io condivido a pieno;

Compagna. Il turismo culturale è infatti - e sempre più deve essere - elemento trainante del settore. Vedo pertanto un'armonia di funzioni nell'attuale assetto del Ministero,

e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». È un unico articolo e, quindi, il riferimento all'attuale organizzazione del Ministero mi sembra assolutamente utile. Il senatore Panizza ha parlato a lungo condividendo l'impostazione del provvedimento

di dare dignità alla retribuzione nel mondo del lavoro, con un intervento importante. Tutta la Commissione è stata molto sensibile a questo aspetto e la delega prevista sarà molto importante. Condivido la preoccupazione e anche la sollecitazione della senatrice Blundo

in questo settore. Ma accanto, ben vengano anche risorse private che, giustamente, come in molte altre parti del mondo, già rappresentano una parte importantissima del finanziamento. In questo senso, abbiamo proposto non solo l'estensione dell'Art bonus, ma anche la valorizzazione dell'associazionismo e il collegamento con il terzo settore (ossia con tutti quei soggetti che possono incrementare questo mondo e anche i finanziamenti e le risorse destinate al mondo della cultura).

pubblica realizzi un impatto culturale e territoriale nel migliore dei modi. Questa riforma, quindi, tende a creare le premesse per un approccio di sinergia e leale collaborazione, l'unico - a mio avviso - che possa creare

è stata protagonista del lavoro di Commissione con le sue proposte, con i molti emendamenti su cui abbiamo discusso.

sempre tutto soltanto sulle fondazioni lirico-sinfoniche forse non è nemmeno sbagliato, ma voglio rispondere sulle questioni delle fondazioni. fondazioni. La lettura del disegno di legge impone una riflessione su come in effetti i problemi non siano molto cambiati prima e dopo la trasformazione in fondazioni con natura giuridica di diritto privato, era uno degli elementi della riforma Veltroni di cui la senatrice ha parlato. E questo ci aiuta a focalizzare le strategie su un approccio un approccio totalmente diverso: rimettere in discussione nuovamente il modello potrebbe avere un costo elevato e non essere risolutivo. Non possiamo adesso tornare indietro e pensare di ripubblicizzare completamente le fondazioni dopo tutti gli anni in cui le stesse hanno fatto

uno dei nodi che il Ministro ha ben presente e vedremo come risolverlo. Nessun intento persecutorio si ha, quindi, nei confronti delle fondazioni; nessuna volontà di interferire nella loro progettualità tagliando risorse. Vi è, invece, una forte volontà di richiamare gli organi di gestione alla responsabilità e al rigore negli investimenti, che è ciò che talvolta è mancato. Tutto questo produrrà non certo un decadimento e si pone come condizione necessaria per un rilancio. La crisi dei corpi di ballo, su cui diversi senatori sono intervenuti, e di cui tanto abbiamo parlato in Commissione e che ci stanno molto a cuore, indubbiamente deriva da una situazione complessiva poco sostenibile, che purtroppo ha condotto a scelte a radicali da parte di alcune gestioni di fondazioni. Confido che una nuova impostazione possa aiutare a riconsiderare all'interno delle varie fondazioni tali scelte, forse a suo tempo obbligate, e ricordiamo dei soggetti significativi che lo hanno voluto. Riguardo all'impegno del Governo sulla cultura, mi pare incontrovertibile che ci siano stati investimenti che da anni non si facevano sia su questo settore - abbiamo reintegrato i bilanci delle fondazioni più volte in questo quinquennio - che sul personale non tanto delle fondazioni quanto più in generale del Ministero, naturalmente con una certa fatica, ma con una prospettiva che non può che far pensare a uno sviluppo complessivo. Il senatore Marin, molto criticamente,

ovvero predisporre, signor Presidente, un provvedimento organico sullo spettacolo, che portasse a prospettive di sviluppo del settore, considerando - come dice la senatrice Idem - che la cultura non è un bene di lusso, ma una materia prima di cui non possiamo fare a meno per plasmare il nostro nostro futuro. Usando le parole della senatrice Ferrara, possiamo dire che, in fondo, quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è dare una risposta a quanti credono che il diritto alla cultura e al patrimonio culturale sia un diritto intangibile di tutti i cittadini. Ringrazio quindi la senatrice Ferrara perché

Grazie

larga di quella parlamentare. Io faccio parte di quelli che pensano che quando la maggioranza su un provvedimento riesce ad allargare i propri consensi non è motivo di imbarazzo, ma è motivo di successo

Ho ascoltato bene le preoccupazioni del senatore Giro e vorrei tranquillizzarlo: non mi sogno e non mi sognerò mai di fare un paragone (anche perché non bisogna mai farlo in prima persona) tra quello che ha fatto questo Governo, o i due Governi in cui ho fatto il Ministro dei beni e delle attività culturali, e i precedenti. Ogni provvedimento è frutto del lavoro degli altri, compreso il fatto che alcuni incentivi, come l'Art bonus, sono stati inseriti nel nostro ordinamento dopo che sono state fatte numerose battaglie da Governi precedenti di diverso colore.

uno sgarbo nei confronti dell'Assemblea, ma ero a Corfù in una bilaterale Italia-Grecia con il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri e numerosi altri Ministri esattamente quella mattina e una parte di quell'incontro bilaterale era dedicato ai temi della cultura. Ho ascoltato le preoccupazioni che sono state espresse - mi fermo a quelle che in parte sono state riprese dalla relatrice - rispetto a un tema che ha sollevato molto dibattito, dal senatore Giovanardi ad altri, che si sono preoccupati del futuro dei circhi. È un tema ben chiaro e dobbiamo avere la consapevolezza di operare per tutelare il futuro della grande tradizione italiana dei circhi, conciliandolo con una sensibilità che via via è cambiata. Non è un problema di condizioni estreme; è una sensibilità che è cambiata profondamente negli anni e anche dagli anni, senatore Giovanardi, in cui da bambini andavamo nei circhi. Rispetto al tema della tutela

soluzione utile e sensata che consenta di rispettare la nuova sensibilità nei confronti del tema della tutela degli animali che, come lei sa bene, è molto trasversale. Non appartiene a uno dei tre schieramenti; è molto trasversale, come lo è il dovere di salvare la grande tradizione dei nostri circhi.

consente di non irrigidire le norme in una situazione sempre in evoluzione. Non è una presa di potere da parte del Ministero o del Ministro, tanto più che ci sono le elezioni politiche all'inizio del prossimo anno e, quindi, vedremo chi le vincerà, che Governo si formerà e chi sarà Ministro. Quindi, non sarà sicuramente questo Governo o questo Ministro

a settori nuovi come la musica popolare e contemporanea e - su richiesta parlamentare - i carnevali e le rievocazioni storiche, tutti settori che non c'erano nel precedente FUS. Come è stato fatto dal Parlamento nella legge sul cinema, il 3 per cento viene destinato all'attività formativa e, quindi, alle scuole.

piacere l'Assemblea che ormai siamo arrivati a circa 180 milioni di euro di donazioni e a oltre 3.500 donatori tra imprese e privati. L'Art bonus è stato introdotto nel nostro ordinamento come misura temporanea

ai teatri di tradizione. In questo provvedimento si adotta una misura sacrosanta perché non aveva senso che utilizzasse l'Art bonus e, quindi, il contributo di privati con un'agevolazione fiscale chi si occupava di musica sinfonica o di lirica e non invece chi fa teatro o prosa. Con il provvedimento viene esteso alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, ai festival alle imprese e ai centri di produzione teatrale di danza, ai circuiti di distribuzione senza scopo di lucro che svolgono attività nel settore dello spettacolo. È un modo forte di aiutare perché l'aiuto è in forma diretta attraverso il FUS e in forma indiretta incentivando

molto tranquilla, vorrei capire perché si eliminano dai circhi, sia pure in maniera graduale, tutti gli animali (compresi i cani e i cavalli), ma non mi sembra che essi vengano eliminati dal cinema

a salvare gli esseri umani sono gli animali appositamente addestrati, anche con grande rigore, per salvare vite umane. Se dovessi portare fino all'estremo limite questo ragionamento, non potrei addestrare gli animali per quelle finalità ciò mi sembra un atteggiamento animalista "talebano", che non ha nessuna giustificazione e che non è neanche di amicizia verso gli animali. Signor ministro Franceschini,

verrà approvata la norma in esame, non avrà più senso. Dice infatti la preghiera dei circensi: «Noi ti ringraziamo, nostro buon Protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa' che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi» La preghiera dice persino: «Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa' che avvenga dopo lo spettacolo e, in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini». se non è collaborazione, se non è amicizia, se non è lavoro comune la preghiera di un *clown* che dice: «In caso di disgrazia, salva prima gli animali, piuttosto che salvare noi». «Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa' che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore». Caro Ministro,

Tutti gli esperimenti di circhi senza animali sono falliti, perché i bambini, come i miei nipotini, che vanno a vedere il circo, aspettano di vedere gli animali, ovvero quello che hanno visto solo in televisione, non potendo magari andare ai safari in Africa.

con i nipotini ho visto uno che faceva la pantomima di Zorro mentre combatte a cavallo contro le guardie. Con questa norma, dentro il circo, nessuno può più presentarsi a cavallo di un animale, perché sarà proibito. Se le cose devono essere fatte in maniera razionale, qualcuno mi deve spiegare perché questo provvedimento è così punitivo e così denso di cattiveria verso un settore che così tanto ha dato all'Italia e che è così famoso nel mondo.

Ebbene, io non voglio che questa tradizione, questa cultura, queste donne, questi uomini e questi artisti muoiano. Io voglio che continuino la loro attività, naturalmente con una grandissima attenzione al benessere animale: controlli, controlli, controlli e ancora più controlli!

L'eliminazione, no. Ripeto, infatti, che: o si e conseguenti e si elimina l'utilizzo degli animali da ogni forma di spettacolo e di presenza nella nostra società; oppure, non si può fare l'eccezione solo per i lavoratori del circo. Ella ha poi detto, giustamente, che vi è una sensibilità.

Ma noi facciamo studiare i bambini, "i cuccioli di uomo", vanno a scuola; che un cane venga addestrato a salvare gli uomini dai terremoti e dalle valanghe, vivaddio, mi sembra una cosa assolutamente giusta e necessaria.

intendo illustrare l'emendamento 1.225

che dovrebbero ispirare l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo (e anche della loro promozione), promozione), il principio che vi siano delle attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività. e l'attività. Riteniamo che inserire espressamente questo principio nel testo del codice sia superfluo oltre che pericoloso. Superfluo perché, in realtà, queste attività sono già consentite a discrezione del sovrintendente, quindi, non capiamo l'utilità di inserire un passaggio ridondante che, anzi, potrebbe avere dei risvolti pericolosi, in quanto potremmo poi trovarci di fronte a delle attività Grazie

sensibilità, anche perché ha sostenuto in pieno le ragioni dell'emendamento e quindi mi auguro che il Governo, che pure ci ha costretto a ritirare gli emendamenti, possa accogliere l'impegno, a ripristinare le agevolazioni del 2 per mille ma soprattutto estendere finalmente anche alle associazioni culturali la possibilità di detrarre parte delle spese per i corsi di formazione e tutta una serie di

2, che vengono tutti proiettati verso lo stesso risultato, su cui si è aperta una dialettica parlamentare che, come tutte le dialettiche parlamentari importanti, verte su cosa vogliamo fare di questo provvedimento.

che alcune specie animali, specialmente quelle su cui verte la polemica (gli elefanti e gli animali selvatici), vengano eliminate. La nostra preoccupazione concerne quel minimo di presenza scenica data, ad esempio, dai cani e dai cavalli,

o anche di superamento dell'utilizzo di alcune specie animali. Il Governo, nella legge delega, scriverà che gli animali selvatici, gli elefanti e tutta una serie di animali che non vengono utilizzati normalmente, non siano più utilizzati, ma non darà questa condanna totale al circo, immotivata e incomprensibile. Vorrei che qualcuno dei colleghi mi spiegasse perché,

Signor Presidente, per un certo verso mi scuso, ma per un altro verso sono contento che la dialettica parlamentare consenta eventualmente di progredire nella ricerca di un

legge si utilizza l'espressione «graduale eliminazione», che vuol dire che ogni specie animale in futuro non potrà essere utilizzata nei circhi equestri. Sollevavo prima il problema non secondario che il circo equestre è nato come circo con i cavalli. Basta guardare la grande pittura impressionista francese per sapere che cosa sia il circo con i cavalli, che però, sulla base di questa norma, dovrebbe

allora ci può stare bene anche il graduale superamento. Però bisogna che lo si dica, perché se «superamento» è uguale a «eliminazione», non caviamo un ragno dal buco. Se invece il superamento è un'indicazione per arrivare ad eliminare gli animali che la sensibilità popolare oggi non ritiene più utilizzabili nei circhi, ma mantenendo quegli animali che lavorano e collaborano ovunque con l'uomo, questo potrebbe essere un compromesso accettabile per noi, ma anche per i lavoratori dei circhi. Signori, io voglio bene agli animali, però vorrei che questa Assemblea ricordasse qualche volta che, oltre ai diritti degli animali, ci sono anche i diritti dei lavoratori: 8.000 lavoratori che rischiano di perdere il posto sono un problema sociale molto rilevante, perché si perde anche il patrimonio di conoscenze di questi lavoratori e la loro capacità artistica. Se il Governo si esprime in questa maniera, potremmo anche arrivare - ma bisogna che il relatore presenti un subemendamento - a ritirare i nostri emendamenti.

in particolare chiede di prevedere delle misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi. In merito alla questione ci sono stati incontri pubblici e dibattiti, all'interno dei quali è emersa la possibilità di avere dei *software*, che sono al momento utilizzati, ad esempio, da una società di Modena, per la

per esempio, non si prevede una sorta di Daspo per i sovrintendenti che nel corso degli anni hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire le fondazioni lirico-sinfoniche. Non faccio i nomi in quest'Aula, ma chi è del settore sa benissimo che mi riferisco ai soliti noti che, per nomina ministeriale, vanno ad occupare il posto di sovrintendente con un giro di valzer da una fondazione all'altra, passando, per esempio, da Bari a Roma o da Roma a Verona.

è stato deleterio per la gestione delle fondazioni ed esprimere parere favorevole - la stessa preghiera la rivolgo alla relatrice - all'emendamento 2.206 che prevede delle misure semplicissime, che non abbiamo inventato noi, ma che rispondono a richieste che arrivano da chi vive il mondo delle fondazioni lirico-sinfoniche in tutti i suoi settori. meno la nomina dei sovrintendenti, selezionandoli invece con bandi pubblici, anche internazionali, permettendo la consultazione pubblica del *curriculum* dell'aspirante candidato. inoltre l'assenza di interessi di qualsiasi natura per tutte le cariche apicali. Quando il Ministro avrà

è lasciati liberi di andare a svolgere attività altrove. Credo che questo sia il minimo sindacale indispensabile per dare un messaggio di serietà a chi vive in quel mondo, che oggi sta pagando. Infatti, c'è da dire che chi oggi sta pagando la *mala gestio* nelle fondazioni non sono gli organi apicali, non è

di un'altra cosa. sovrintendente che sale sul palco come *one man show*. Quindi, signor Ministro, la prego veramente di riflettere su questo. Noi le stiamo dando una grande opportunità con questo emendamento.

ma tanto vale riflettere per lasciare ai posteri una buona indicazione.

- dà l'indicazione di questo passaggio anche culturale di riconversione che è nell'interesse dei circhi e delle attività circensi. Abbiamo esempi, in altre parte del mondo, di spettacoli circensi bellissimi, che anche nel nostro Paese

Mi taccio facendo un ultimo appello: questo è un elemento importante e forte per avviare una riconversione; il Ministro deve stare tranquillo perché è in sintonia con l'opinione pubblica, con la nuova sensibilità maturata in questi anni. Soprattutto questo servirà a salvare il circo; diversamente non si agisce certamente nell'interesse di questa antica tradizione.

Visto che la relatrice ha riconosciuto con la sua proposta di riformulazione che, in effetti, l'emendamento può essere suddiviso in due parti, chiedo se è possibile procedere alla votazione per parti separate.

Il problema è che il voto per parti separate dovrebbe far sì che, se una parte viene approvata e l'altra no, abbia comunque una sua autonomia e sia comprensibile da un punto di vista letterale.

questi contenuti li abbiamo già previsti in altre parti del disegno di legge. È, infatti, detto espressamente che le attività di spettacolo debbano avere uno spazio specifico all'interno della programmazione RAI.

è l'attivazione del tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Ente nazionale italiano per il turismo proprio per la valorizzazione, attraverso i percorsi di arte, dello attraverso i percorsi di arte, dello spettacolo che può servire in questo senso. Visto che la prima parte è già ampiamente trattata e introdotta nel provvedimento, mi sembra francamente abbastanza inutile votare per parti separate,

Grazie

in questo caso il Governo e la relatrice abbiano perso una grande occasione per iniziare a sanare questa situazione, che - lo ribadisco - prima o poi, come un nodo, arriverà al pettine. Anche in questi giorni se ne sta parlando e

si è inventato di sana pianta tale necessità, ma anche l'Autorità *antitrust* ha aperto una procedura di indagine rispetto alle attività della SIAE, a seguito delle numerose segnalazioni che ha ricevuto dagli artisti e dagli utilizzatori. Quindi, anche questa volta mettete la testa sotto la sabbia, ma il problema si ripresenterà.

una veloce dichiarazione di voto su questo emendamento perché, nonostante l'occasione che abbiamo dato, sia al Ministro che alla relatrice e, quindi, anche alla maggioranza e al Governo, di fare una cosa buona per le fondazione lirico-sinfoniche, per il loro futuro e per la loro gestione, questa occasione è stata rifiutata. Leggiamo, allora, cosa hanno rifiutato. Esprimendo un parere contrario a questo emendamento e votando

probabilmente, a essere sottoposti a delle logiche più politiche che di merito: continua ad esserci questo grave pericolo. Continuerà ad esserci questo pericolo e, forse, continueranno ad esistere, all'interno di alcune fondazioni, conflitti di interesse fra sovrintendenti, direttori artistici o, comunque, organi apicali che possono avere cotitolarità all'interno di agenzie teatrali e, quindi, decidere quali artisti lavorano, o non lavorano, non in base a logiche di merito, ma in base a logiche di profitto o clientelari. continueremo ad assistere al valzer delle stagioni dei sovrintendenti che si sono distinti per la *mala gestio* delle fondazioni e che continueranno a danzare tra una fondazione e l'altra. questa loro *mala gestio*, continueranno a pagare soprattutto (anzi, esclusivamente) le masse artistiche e tecniche.

tra i criteri per l'erogazione dei fondi ci sarà l'eventuale individuazione della responsabilizzazione del sovrintendente nella gestione, che è il massimo che siamo riusciti ad ottenere.

ci saranno altri incontri con gli operatori delle fondazioni lirico-sinfoniche, questo fatto le sarà ampiamente ricordato. Lei sta perdendo una grande occasione, dimostrando una profonda incapacità di ascolto.

la seconda parte, cioè sul punto 3) in cui si legge: «nei casi di casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al soprintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni»,

pone un tema puntuale rispetto a tutto il disegno di legge, che è il rapporto tra pubblico e privato. Il ministro Franceschini, nel suo intervento in replica, ci ha riferito che con l'Art bonus sono stati raccolti oltre 180 milioni di euro. euro. Con questo emendamento vogliamo dire che l'intervento di finanziamenti privati non può assolutamente costituire un alibi per eliminare l'investimento che deve necessariamente fare il pubblico,

infatti, abbiamo detto che i tagli profondi alla cultura hanno portato in questi anni a un impoverimento culturale dell'intero Paese e pensare di dover sostituire l'investimento e il ruolo del pubblico con il ruolo del privato vorrebbe dire non aver assolutamente risolto il problema.

di circa 13 metri creata per permettere l'esibizione armonica dei cavalli che ne costituiscono il fondamento. Quindi, nella tradizione del circo equestre italiano, esso è costruito per far esibire i cavalli. È evidente che l'eliminazione di ogni tipo di animale dal circo vuol dire semplicemente cancellare la tradizione del circo italiano e la sua storia. Pensate soltanto alle decine di film,

che hanno tutto il diritto di esistere. Tuttavia, davanti ad obiezioni ragionevoli (che comunque fanno fare un passo avanti nella loro direzione rispetto a determinate specie animali), tali

che non sono proibite, anzi vengono agevolate dallo Stato, come quelle che ho ricordato prima. Pertanto, chiedo se sia possibile, per una questione di stile e di forma, non votare questo emendamento ed accantonarlo, mettendolo nel sacco con gli altri.

a risolvere il problema cui si è fatto cenno in precedenza con riferimento ad un emendamento presentato dalla senatrice Montevecchi, sulla strada dell'armonizzazione dell'ordinamento italiano in materia di tutela di diritti d'autore rispetto alla direttiva europea.

una scappatoia nei confronti della norma che prevede il progressivo abbandono dell'utilizzo degli animali nei circhi, con un gioco semantico,

poiché il legislatore ha manifestato chiaramente la volontà che in Italia si vada verso la progressiva dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi, credo

di avanzamento su un terreno difficile, delicato e fragile dell'umanità, della natura e del rapporto tra l'uomo e la natura, anche attraverso tutti quegli esseri viventi che sono gli animali.

non tanto e non solo con una questione culturale, ma anche con una questione molto più terrena, che attiene non solo alla cultura, ma proprio al rispetto di noi e di tutti gli esseri senzienti.

Penso che quando è in ballo il divertimento dell'uomo, il tempo non possa essere fermato. Ma quel divertimento, se passa attraverso la sofferenza di un altro essere, per me non è più tale.

Concludo questo mio breve intervento, che è solo una dichiarazione di voto a sostegno dell'istanza di un nuovo rispetto nei confronti degli animali, anche attraverso la modalità degli spettacoli viaggianti, del circo e del divertimento in generale, ovunque ovunque questo si realizzi (su questo ha ragione il collega Giovanardi). Concludo ricordando al collega Giovanardi e a tutti coloro che si ispirano anche a importanti culture e tradizioni religiose, che «anche gli animali sono creature di Dio, che nella loro muta sofferenza sono un segno dell'impronta universale del peccato e dell'universale

fare cultura e spettacolo con lo sfruttamento degli animali non ci porta da nessuna parte. Abbiamo la possibilità di far vedere ai nostri figli gli animali in libertà attraverso migliaia di possibilità (penso a tanti canali televisivi, anche specifici, che entrano nelle nostre case tutti i giorni). Vi ricordo, colleghi, che l'unico circo del mondo in attivo che viene in tutte le città d'Italia, tra cui Roma, che fa *overbooking* di biglietteria e non riesce a soddisfare tutte le prenotazioni è il Cirque du Soleil, un circo nel quale esistono solo umani. Ebbene, io penso che l'uomo debba stupire l'uomo con le sue capacità: non c'è una tigre che salta nel fuoco che mi stupisce più di un trapezista o di un giocoliere o comunque

capitano quei grandi camion, dove dentro c'è uno squalo o una tartaruga d'acqua, che si appostano nelle grandi periferie delle nostre città chiedendo un biglietto ridicolo, di uno, due, cinque euro, per tenere quell'animale in una sofferenza perenne. Mi domando, allora, perché noi che stiamo discutendo di un immenso cambiamento, finalmente con un nuovo regolamento, non vogliamo mantenere la barra dritta su ciò su ciò che nel mondo è ormai in via di superamento. Hanno parlato alcune colleghe prima di me, ma io vi dico che anche i nostri sindaci sono in grande difficoltà: ci sono decine di sindaci che non concedono più l'occupazione di suolo, che non danno le aree ai circhi che hanno animali. Poi ci sono i ricorsi al TAR. Pertanto, veniamo incontro a chi fa uno sforzo eliminando gli animali dal suo spettacolo, facendo, per esempio, una politica di incentivazione fiscale, prevedendo alcuni sgravi, concedendogli gratuitamente le aree nei Comuni a fronte della dismissione degli animali. Allora sì, signor Ministro, potremmo mantenere un supporto e un aiuto ai circhi che, rinunciando allo sfruttamento, all'ostentazione degli animali in cattività, mantengono la parte preponderante del loro spettacolo dove è l'uomo che stupisce, l'uomo con le sue capacità. Questo potrebbe incentivare e non abolire una tradizione circense, che è quella, per esempio, della grande scuola di Verona, dove i nostri giovani imparano a diventare trapezisti piuttosto che giocolieri o acrobati. Proviamo in questo modo a mantenere una tradizione con un aiuto concreto, ma diamo finalmente un segnale e allineamoci all'Europa. Colleghi, i bambini capiscono che la tigre che salta nel fuoco non lo farebbe mai per sua libera scelta, e se dobbiamo fare cultura facciamola veramente.

domanda: il benessere animale vuol dire essere tutti schierati contro ogni forma di sfruttamento o di attività che porti sofferenza agli animali? Sì, su questo non ci piove. però, sosteniamo che l'utilizzo degli animali in qualsiasi forma è sfruttamento, allora, ripeto, perché con un provvedimento come questo o con un provvedimento analogo non proibiamo l'ippica? Gli ippodromi devono essere chiusi o devono rimanere aperti? Alle olimpiadi le attività ippiche, il *dressage* devono essere fatti o è sfruttamento del cavallo? In tutte le attività del cinema e del teatro in cui vengano utilizzati gli animali questo è possibile o deve essere proibito? Il Palio di Siena deve continuare o essere abrogato? Io conosco la risposta delle colleghe che sono intervenute prima di me: tutte queste cose devono essere eliminate.

quando dal quinto piano scende il cane vestito in un certo modo o che comunque viene utilizzato dalla signora anziana come compagnia, quel cane non sta svolgendo una funzione relativa alla sua natura, ma sta facendo un servizio a quella signora ed io lo ritengo anche giusto, perché non ritengo che le persone non possano tenere un cane nell'appartamento, anche se in realtà, riparametrando il discorso che facciamo sui circhi, come il cane non può lavorare nel circo, allo stesso modo non potrebbe stare neanche in un appartamento. Se vogliamo ottenere

compromesso onorevole, che soprattutto non ci copra di ridicolo davanti al mondo, perché in Europa non c'è Paese dove non si possano utilizzare gli animali.

Parliamoci chiaro: questo è un processo di riconversione che non pone soltanto la questione del rispetto degli animali, che non possono essere utilizzati per il nostro divertimento. Ma cosa c'entrano gli animali di affezione con il loro utilizzo a fini di spettacolo?

le prenotazioni per soddisfare tutte le richieste) un grande circo come le Cirque du soleil, che è fatto di grandissimi artisti: acrobati, giocolieri e una scuola che ha reso di nuovo viva e importante

attuano diversità di trattamento. Faccio un esempio: il cavallo e il mulo che vengono utilizzati in montagna per trasportare la legna in luoghi impraticabili sono sottoposti a fatica e a stress? Oppure lo fanno per divertimento? Lo stesso vale per il cavallo o altro animale che viene impegnato in un spettacolo. Un delfino che viene incentivato a saltare continuamente, lavorando e producendo spettacolo, è nel massimo della sua esaltazione di libertà, oppure anche lui viene orientato rispetto a certe fatiche? Credo che dobbiamo approcciare il problema con minore radicalità, sapendo che c'è un'evoluzione che non è necessaria di indurre per legge, ma passa attraverso una maturazione culturale. Non vedo la necessità di imporre percorsi obbligati e vietare in assoluto determinati utilizzi, perché

che tra un uomo e una patata c'è un po' di differenza. alle osservazioni già espresse dalle colleghe, in particolare dalla collega De Petris, volevo aggiungere una domanda. Si chiede l'accantonamento di due emendamenti

intervengono sulla lettera *h)* aggiungendo le parole: «e di spettacolo viaggiante» dopo le parole in tema di «attività circensi». Vorrei chiedere alla Presidenza, alla relatrice e al Governo di valutare quale attinenza possa esservi tra questi due emendamenti e quelli proposti dal senatore Giovanardi, perché effettivamente i nostri intervengono sulla lettera *h)*, mentre quelli del senatore Giovanardi sulla lettera *o).* Credo non ci sia nessuna connessione logica tra gli emendamenti del senatore Giovanardi e i nostri, che hanno come obiettivo del senatore Giovanardi intervengono su altra materia, seppur affine perché parliamo sempre di utilizzo di animali presenti nei circhi. Aspetto una risposta. *(Applausi

a trovare una conciliazione su un elemento. Non si può passare improvvisamente da una situazione che, tra le altre cose, è radicata nella tradizione a una situazione completamente opposta. Per arrivare a fare il circo 4.0, 4.0, bisogna fare il circo 2.0, 3.0 e poi si arriverà al 4.0. Mi sembra di aver colto nell'intervento del ministro Franceschini una consapevolezza importante in questo senso, perché dire che c'è bisogno di una soppressione graduale, a mio modo di vedere, significa due cose: non solo che la gradualità va interpretata nel tempo, ma anche rispetto alle diverse specie di animali. È chiaro che ve ne sono alcune per cui i maltrattamenti

intervengo solo per richiamare l'attenzione sul fatto che la senatrice Montevecchi ha ritenuto di fermarsi alla questione della lettera *o)-bis* degli emendamenti presentati

vorrei ricordare che ormai da decenni non vengono più presi animali selvatici nelle foreste o nelle savane; la riproduzione degli animali avviene direttamente nei circhi. Sicuramente, quegli animali potranno mai essere ricollocati, né

vorrei sottolineare un aspetto che ho già evidenziato nel mio intervento in discussione generale. L'intervento del senatore Giovanardi mi ha creato grande sofferenza e continuano a procurarmi grande sofferenza anche gli interventi di oggi e i paragoni effettuati.

non tengono gli animali nelle dovute condizioni. Credo, però, di non essere l'unica a vivere in una città di provincia che vede certi fenomeni. Voglio anche ricordare che la questione dello spettacolo viaggiante è già nella sfera del MIBACT. Quindi, bene hanno fatto le colleghe e i colleghi

questione non solo di civiltà ma anche economica. E non è vero, senatore Ranucci, che il Cirque du Soleil va solo a Las Vegas. Abito a Viareggio e per fortuna, grazie alla illuminata

E lo possiamo fare calendarizzando un disegno di legge sollecitato da più di due anni da milioni e milioni di persone.

Signor Presidente, la discussione che si è instaurata oggi ha una portata molto ampia e non riguarda solo il benessere degli animali dei circhi viaggianti e dei circhi equestri.

basta andare a vedere la fine che fanno i cavalli quando non corrono più nei galoppatoi: vengono mandati sistematicamente al macello.

sarà chiamato a svolgere le funzioni particolarmente importanti per il settore dello spettacolo dal vivo, perché esprimerà pareri, darà le linee guida al Ministero, formulerà delle proposte e guiderà anche dei tavoli tecnici, credo che sarebbe opportuno, come un gesto minimo sindacale, rendere pubbliche le sue attività, soprattutto in riferimento ai pareri o agli atti inerenti lo stanziamento o la gestione delle risorse pubbliche. Mi auguro che sull'articolo 3 ci sia un buon ascolto e si prenda spunto dalle proposte emendative che arrivano dal Movimento 5 Stelle, perché questa potrebbe essere un'occasione per iniziare a introdurre le nuove prassi, un nuovo *modus operandi* all'interno dei consigli superiori. si chiede di dare maggiore trasparenza alle attività, anche perché ricordo che quelli pubblici sono soldi dei cittadini e, quindi, è giusto che un qualunque cittadino abbia la possibilità, qualora interessato, di verificare le attività di controllo e monitoraggio del consiglio superiore.

si debba garantire la maggiore rappresentatività possibile nel perimetro dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività del consiglio

a livello decisionale quando ci sarà da controllare, monitorare e proporre anche sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si è data la

Signor Presidente, intervengo in merito alle gravi e sconcertanti dichiarazioni fatte il 15 settembre scorso dal senatore D'Anna in un'intervista a Radio Cusano Mi limiterò a citare qualche dato per ricordare la portata dell'assurdità delle affermazioni di un membro di questo Parlamento.

ricordare che ci sono 6 milioni di vittime in Italia. Il 21 per cento delle donne italiane, pari a 4,5 milioni, è stato costretto a compiere

«Sono abbastanza vecchio per ricordarmi donne più accorte. Una donna aggredita da un cingalese alle 3 di mattina un tempo non ci sarebbe mai stata. La donna porta con sé l'idea del corpo, l'idea della preda. Se si trova in una zona di periferia sola, in mezzo alla strada, può anche essere oggetto di un'aggressione. Se cammina un uomo solo alle 3 di notte, non gli succede niente. Se cammina una bella ragazza, magari vestita in modo provocante e si trova in determinati ambienti, si espone. Qui tutti vogliono fare tutto. Io non sono un maschilista, ma il corpo della donna è oggetto e fonte di desiderio da parte dell'uomo. È un istinto, sarà primordiale, ancestrale, quello che volete. Molte volte servirebbe un minimo di cautela. Le donne devono pensare che c'è gente in giro che può far loro del male. Le donne hanno un *appeal* diverso da quello degli uomini. Potrei parlare degli ormoni, dell'aggressività. Certe volte volte un tipo di abbigliamento, un tipo di contesto fa pensare a dei soggetti che siano una manifestazione di disponibilità da parte della donna. Serve un po' di buon senso, un poco di cautela, alle donne non farebbe male. Non è una manifestazione di inferiorità». No,

bisognerebbe escludere gli animali che qua dentro sono presenti, che a tutto titolo devono essere considerati una razza inferiore. Il senatore D'Anna si deve vergognare. E parimenti devono vergognarsi il presidente Grasso e la presidente Boldrini,

la staffetta con cui, insieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo sino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al Paese tutto l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Sono ad oggi 79 le donne che abbiamo ricordato e, dal 2 luglio, data del nostro ultimo intervento, sono state uccise altre 10 donne. Le ricordo:

anni, è stata strangolata dal suo fidanzato, che ha poi vagato tutta la notte con il suo corpo accasciato sul sedile del passeggero. Il 4 agosto a Ferrara, Mariella Mangolini, di settantasette anni, è stata uccisa con un colpo di pistola dal marito, che ha poi ucciso allo stesso modo il figlio di Il 17 agosto, a Dogaletto di Mira, in provincia di Venezia, Sabrina Panzonato, di cinquantadue anni, dopo essere stata ferita con una coltellata al fianco, è fuggita in strada, dove l'ha raggiunta il marito e l'ha uccisa con un colpo alla testa, per poi suicidarsi. La coppia lascia soli due figli.

per ustioni gravi su tutto il corpo. Ma non si trattava di un incidente domestico: il 6 settembre il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio, per avere dato fuoco volontariamente alla moglie, come ultimo atto di una lunga serie di maltrattamenti e violenze nei suoi confronti. Decisiva è stata la testimonianza del figlio di dieci anni. Il 3 settembre, a Specchia, in provincia di Lecce, Noemi Durini, di sedici anni, è stata uccisa dal fidanzato di diciassette anni. Il ragazzo era stato denunciato alla procura dalla mamma di Noemi per violenze nei confronti della figlia. Erano, infatti, in atto due procedimenti, uno penale e uno civile, nei suoi confronti. L'8 settembre, il gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato l'arresto dell'ex fidanzato di Alessandra Madonna, di ventiquattro anni, accusato di averne provocato la morte, trascinandola con l'auto nel parco in cui risiede, a Mugnano di Napoli. Il 9 settembre a Donoratico, in provincia di Cagliari, Joelle Demontis, di cinquantotto anni, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. La donna portava ancora i segni di percosse probabilmente subite nei giorni precedenti la morte. Per l'omicidio sono stati arrestati il compagno della donna e una ragazza di ventisei anni che abitava con loro. Il 15 settembre, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, Elena Seprodi, di quarantotto anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex marito nella sua abitazione al culmine di un litigio. La donna lascia un figlio. Mi sono sempre chiesta cosa succede nella testa di quell'uomo che trasforma quasi in una sagoma di cartone, contro cui scagliare la propria furia omicida, la donna con cui ha condiviso passione, amore, sogni, progetti e magari ha generato figli. ha generato figli. Questa domanda è importante, ma è bene ricordare che noi donne siamo persone, non semplici cose di cui disporre a proprio piacimento. Abbiamo buone leggi: il Governo e il Parlamento, nel corso del tempo, hanno fatto molto e molto stanno facendo. Sto pensando al rafforzamento della rete delle case rifugio, all'introduzione del congedo retribuito per le donne lavoratrici, comprese quelle autonome, quando devono allontanarsi da casa, per la loro sicurezza. Sto pensando all'educazione di genere inserita nella legge sulla buona scuola. E dovremo sicuramente lavorare per fare ancora di più sul versante della certezza della pena. E l'auspicio che faccio è che il Parlamento e il Governo rafforzino, anche nella prossima legge di stabilità,

quindi, sono importanti, ma tutto questo non basta, perché il problema è culturale. Il problema sono quegli uomini, sempre più numerosi, che, non essendo capaci di ritrovare dentro se stessi un nuovo equilibrio, scelgono di uccidere piuttosto che accettare la fine di una relazione amorosa. Il problema sono quelli uomini che di fronte - ad esempio - agli stupri e alle violenze, dicono che le donne devono essere più caute. Quando una relazione amorosa finisce, può aprirsi il baratro dell'abbandono e si deve sicuramente imparare ad andare avanti lo stesso, anche se talvolta può essere doloroso e può sembrare impossibile. Ma tutto questo dolore non può assolutamente giustificare mai la violenza e mai la violenza omicida. È davvero drammatico che tanti uomini oggi non riescano ancora a capirlo né a farsene una ragione, arrogandosi il diritto di strappare alla vita chi da quella relazione vuole uscire. E allora l'impegno e la battaglia sono sicuramente quelli che ho detto prima, ma devono essere anche sul piano culturale ed è su questo piano che dobbiamo lavorare tutti insieme, uomini e donne.

rispettoso all'interno di una relazione, quanto sia bello essere persone libere; amateci per quello che siamo, e cioè persone libere capaci di rispetto anche all'interno di una relazione amorosa. Ditelo, perché l'amore è sicuramente l'energia più potente, ma così, come ci si innamora in modo naturale, è altrettanto naturale e normale che quell'amore sfumi, siano vinti o vincitori. La violenza non è una variante dell'amore: è violenza e basta. Nasce, si sviluppa e si nutre dentro una cultura o sottocultura che ancora oggi ha come contesto lo svantaggio sociale per le donne. Per tutto questo, ripropongo il nostro appello a tutto il Paese e ai *media* dico: smettete di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini. Smettete di chiamarli, come ad esempio in tutte le trasmissioni televisive in cui si parla di Noemi, «il fidanzatino». Non sono fidanzatini o altro: sono assassini. E smettete di colpevolizzare le donne. *(Applausi dai di avere un sussulto, ma non temporaneo, di indignazione e di sdegno permanente, perché sono davvero troppe le donne che vengono uccise. Ormai è una strage che non possiamo più accettare. *(Applausi

che secondo quanto risulta agli interroganti: Isidoro Ferrante è stato condannato per il tentato femminicidio di Lidia Vivoli, episodio consumatosi la notte del 25 giugno 2012 e che ha lasciato sul corpo e nell'anima della Vivoli segni indelebili; il prossimo 10 ottobre 2017 Isidoro Ferrante uscirà dal carcere di Palermo; Ferrante, nonostante le pesantissime accuse di sequestro e tentato omicidio, è stato condannato a soli 4 anni e 6 mesi, in quanto ha usufruito del patteggiamento allargato; dopo 5 mesi di carcere, ha anzi ottenuto i domiciliari, ma li ha evasi regolarmente per pedinare la Vivoli, la quale diveniva così vittima di uno *stalking* assillante, con continui messaggi con i quali l'uomo dimostrava di sapere sempre dove lei si trovasse e cosa facesse; il tutto per due anni interi; pare che Ferrante abbia anche aggredito l'attuale compagno della Vivoli, con cui la donna ha avuto due gemellini di appena un anno e mezzo; nel novembre 2014 Ferrante, incurante del divieto di avvicinamento, affrontava nuovamente Lidia Vivoli, in strada, in pieno giorno, tentando dapprima un approccio e poi colpendola con uno schiaffo che provocava alla donna la lacerazione del labbro inferiore; solo a novembre 2015, a seguito delle nuove denunce, Ferrante è stato condotto nuovamente in carcere,

di muoversi, lei sia costretta a chiudersi in casa, nella sua frazione, per stare al sicuro. C'è poi anche il rischio che il Ferrante non rispetti affatto il divieto, o che trovi altri mezzi per arrivare comunque alla Vivoli o alla sua famiglia, come - sempre secondo quanto sostenuto dalla donna - ha promesso. Ora Lidia Vivoli chiede aiuto e lo fa a gran voce, usando tutti i mezzi di comunicazione, diffondendo anche le immagini che la ritraggono ferita dopo quella notte di giugno. Negli ultimi tempi - come ci ha ricordato prima anche la senatrice Mattesini - è emerso a più riprese come le denunce inascoltate da parte di donne che sono state oggetto di violenza hanno provocato morti ingiuste e laceranti e svelato quanto sia breve il passo dalla minaccia all'epilogo tragico. Occorre evitare in tutti i modi che quello di Lidia Vivoli sia il prossimo caso di femminicidio annunciato. Per questo, assieme ad altri senatori e senatrici del mio Gruppo, ho presentato un'interrogazione per sapere se il Ministro dell'interno sia a conoscenza della situazione di Lidia Vivoli e se ritenga o meno necessario intervenire con urgenza con misure di protezione adeguate e, se sì, quali, a tutela di una donna la cui drammatica vicenda suscita timori più che fondati circa la sua integrità e la sua stessa esistenza. Vorrei quindi chiamare il Parlamento a testimonianza di questa sollecitazione. Presidente, se suo nipote le portasse una pagella dove in *Geschichte* avesse come voto *befriedigend*, lei lo elogerebbe o lo rimprovererebbe? E, se le consegnassero un referto medico con scritto *Ruckenschmerzen*, lei si preoccuperebbe o tirerebbe un sospiro di sollievo? Vede, mentre a lei queste ipotesi possono sembrare assurde, per un padre italiano che ci ha scritto sono la normalità. Sarebbe un fatto normale se parlassimo di un emigrante a Francoforte, ma questo accade su territorio italiano, a Bolzano, dove la scuola alla quale il figlio è iscritto

«Siamo una scuola di madrelingua tedesca e quindi niente italiano né con i bambini né con i genitori italiani. Si può parlare in italiano semmai con i genitori di bambini extracomunitari che, essendo in Alto Adige da poco tempo, non hanno avuto la possibilità di imparare il tedesco»: queste sono parole non raccolte da un avventore al bar, ma di una dirigente scolastica citate dal quotidiano «Alto Adige». E c'è di più:

in risposta l'assessore si raccomandava invece di non esagerare a farlo, come se stesse raccomandando di non esagerare col bere. Se non ricordo male, fu il Presidente Mattarella lo scorso anno a celebrare a Trento l'accordo De Gasperi-Gruber sull'uso paritario della lingua italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni. La tutela delle minoranze linguistiche in Italia va giustamente in difesa dei cittadini di lingua tedesca, ma in Trentino-Alto Adige le minoranze linguistiche da tutelare sono due: l'italiano e il ladino. Chiediamo quindi che sul territorio italiano, dal Brennero a Lampedusa, l'accesso alle informazioni, tanto più se riferite a dati rilevanti come l'andamento scolastico di un figlio o le condizioni di salute di un familiare, debbano essere garantite sempre anche in lingua italiana, ferma restando, sicuramente, la tutela del bilinguismo, come recita la nostra Costituzione.

È una scelta che posso anche non condividere, ma il problema che segnalano i colleghi della Lega Nord è reale: il fatto cioè che, con un provvedimento d'urgenza, tutti i

caso in esame abbiamo un sequestro per una somma enormemente superiore ai fondi di cui sarebbe stato accertato il cattivo uso con una mancanza totale di operatività da parte del partito.

Signor Presidente, ho chiesto la parola, e non ne abuserò, per associarmi alle amare parole del collega Endrizzi, che ancora una volta segnalano una condizione di particolare disagio

a essere una delle realtà più interessanti del nostro Paese; una realtà, però, dove non è possibile tollerare che, partendo da un presupposto di coabitazione, si arrivi invece alla discriminazione quotidiana delle popolazioni italiane residenti in Alto Adige, perché sarebbe davvero un bel effetto paradossale. E, tra le tante situazioni paradossali, quella appena ricordata dal senatore Malan è davvero inquietante, perché agisce direttamente su uno degli strumenti della democrazia previsti dalla Costituzione. Anche la vita delle imprese è segnata da scelte drammatiche, spesso

ma in questo caso va in discussione proprio il sale della democrazia. Quel finanziamento spettava e spetta alla Lega in virtù di una legge dello Stato ed è pubblico, è pubblico, e quelle somme non possono essere oggetto di un abnorme sequestro che nulla ha a che vedere realmente con la sicurezza del fatto che del fatto che debbano essere oggetto di una revisione finanziaria e amministrativa. Lo abbiamo detto già in tante riprese